cari colleghi, signori del Governo, dopo aver abolito in un sol colpo la povertà, oggi Governo e maggioranza compiono un altro prodigio e aboliscono la corruzione. Ci hanno spiegato che, grazie alla cancellazione della prescrizione, che scatterà dopo la sentenza di primo grado, persino se di assoluzione, per i criminali non sarà più possibile sfuggire alla giusta punizione. I perfidi azzeccagarbugli resteranno con un palmo di naso: un efficace *spot* propagandistico, ma un pessimo servizio alla verità, signori della maggioranza e del Governo. È una *fake news*, che ignora dati di fatto incontrovertibili, invano ricordati da più parti anche ieri nel corso della discussione generale, vale che quasi il 60 per cento dei procedimenti penali in realtà si prescrive in istruttoria, mentre un altro 20 per cento entro la definizione del primo grado. Su di essi la riforma non ha ovviamente alcun effetto, ma alla maggioranza e al Governo questo non interessa, è un dettaglio trascurabile e si sa che, quando i dettagli danno fastidio,

vigore nel 2020 e non è retroattiva, perché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale. I reati meno gravi si prescrivono in sette anni e mezzo che, per effetto della riforma Orlando, possono arrivare fino a dieci anni e mezzo. Per i più gravi, come corruzione, peculato e concussione, si arriva a quindici, Se l'aritmetica non è un'opinione, i primi effetti di questa epocale - si fa per dire - riforma, si manifesteranno nel nostro ordinamento giuridico non prima del giugno 2030 e questo solo per i reati meno gravi e comunque al netto delle numerose cause di sospensione della prescrizione, che continueranno ovviamente ad operare nel processo. ci saranno dal 2036, per la concussione dal 2038, per la corruzione tra il 2035 e il 2038, a seconda della gravità della singola fattispecie. La domanda sorge quindi spontanea. Valeva la pena, signori del Governo e della maggioranza, calpestare la Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le fondamenta stesse su cui si fonda da secoli la nostra civiltà giuridica, per una norma che - ammesso ci arrivi, e ho molti dubbi in proposito - produrrà i suoi effetti quando la maggioranza di noi sarà in pensione già da molto tempo, ma che purtroppo da oggi, per una sorta di eterogenesi dei fini, produrrà immediatamente tutti i suoi effetti negativi, trasformandosi nell'alibi con cui sviare l'attenzione da ogni reale stortura del sistema, sia essa organizzativa, gestionale o normativa? Noi crediamo sarebbe stato molto più serio impegnarsi, ad esempio, per studiare come intervenire sui quattro uffici giudiziari in cui si verifica circa la metà di tutte le prescrizioni, vale a dire le corti d'appello di Roma, Napoli, Torino e Venezia, secondo gli stessi dati offerti dal Ministero. studiare come semplificare e snellire la procedura, eliminando formalità ridondanti e superflue, ad esempio, in materia di notifica. Si intervenire anche sulle reali cause delle lungaggini dei processi, che non sono dovute come ci dicono tutte le statistiche, se non in minima parte, all'attività difensiva della quale, signori del Governo, signor Ministro, occorrerebbe maggior rispetto - ma alle carenze degli uffici e degli organici, ai frequenti trasferimenti dei giudici o alle loro assenze, ai difetti o ai vizi di notifica dei testimoni o delle parti ad opera del pubblico ministero e così via. O, ancora, studiare come deflazionare i processi, ampliando il ricorso agli istituti ad esso alternativi, come l'oblazione, il risarcimento quale causa di estinzione del reato, la messa alla prova, l'irrilevanza del fatto, eccetera; o, ancora, operando finalmente una radicale depenalizzazione, magari avendo cura questa volta di non mettere sullo stesso piano chi si appropria di cose di poco valore e chi di milioni di euro, come ha fatto il Governo a guida PD nella scorsa legislatura (ogni riferimento a fatti e persone di cui si è occupata la recente cronaca giudiziaria è puramente voluto); o ancora, per fare solo un ultimo esempio, introducendo in Costituzione la non impugnabilità da parte del pm delle sentenze di assoluzione, in ossequio al principio, che dovrebbe essere sacrosanto in uno Stato di diritto, del ragionevole dubbio. Certo, sono tutte cose più difficili e complicate della facile e illusoria strada che Governo e maggioranza hanno scelto di seguire e di assai minor impatto propagandistico, che in realtà resta il vero scopo di questa norma manifesto. Del resto, parafrasando don Abbondio, si potrebbe dire che il senso di responsabilità uno se non ce l'ha, mica se lo può dare da solo. in esame ci sono anche altre norme, purtroppo di immediata efficacia, che noi non possiamo condividere. Mi riferisco all'articolo 6 che, attraverso le mentite spoglie dell'agente sotto copertura, introduce di fatto la non punibilità dell'agente provocatore, prevedendo addirittura che possa compiere attività prodromiche o strumentali e persino che possa offrire al pubblico ufficiale denaro o qualsiasi altra utilità all'evidente fine di indurlo in tentazione. quindi, di un'attività volta a prevenire e acquisire le prove dei reati, su cui saremmo pienamente concordi, ma a provocarli che, al contrario, si traduce in un altro gravissimo *vulnus* per lo stato di diritto, dalle conseguenze che temo saranno devastanti.

la soglia di pubblicità dei finanziamenti ai partiti, mentre dall'altro alla Camera respinge un emendamento - condiviso anche da Fratelli d'Italia - inizialmente presentato dalla Lega e poi sparito, come molti altri, nella nebbia del compromesso al ribasso. Mi riferisco alla proposta che avrebbe esteso anche alla piattaforma Rousseau le regole di trasparenza dei partiti e delle loro fondazioni. In conclusione, cari colleghi, Fratelli d'Italia avrebbe voluto confrontarsi in quest'Aula nel merito, non solo per tentare di migliorare il provvedimento su questi punti appena illustrati, ma per valorizzare anche quanto di positivo contiene.

le intenzioni del provvedimento in esame sono positive e condivisibili, ma il modo con cui vengono declinate lascia diverse perplessità. La corruzione è un male profondo che penalizza i migliori e gli onesti e distorce le regole del vivere civile. Bisognava continuare sulla strada delle riforme per affermare la piena certezza del diritto, la cui assenza è uno dei problemi più gravi per lo sviluppo del Paese. Si calcola infatti che la lentezza della giustizia costi un punto di PIL all'anno e sappiamo tutti che costituisce uno dei principali ostacoli nell'attrarre investimenti stranieri. Con il provvedimento in esame, però, si è scelta una scorciatoia. Lo si fa, come al solito, per ragioni propagandistiche, per la necessità di mettere una bandierina rispetto alla domanda di maggiore giustizia che viene dall'opinione pubblica, ma lasciando sul tavolo tutta una serie di problemi. Questo vale soprattutto per la prescrizione. Sono d'accordo con la necessità di sospenderla, anche con l'inizio del processo penale, come accade in tanti altri Paesi europei. Non sono pochi i casi dove la difesa punta al raggiungimento della prescrizione e non all'assoluzione dell'imputato. Ma la sospensione della prescrizione, per avere senso, deve essere inserita in una rivisitazione complessiva del processo, mentre con questo provvedimento si aumenta soltanto il rischio di ledere il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Per questo, prima di prima di eliminare la prescrizione, si doveva semplificare il processo penale e riformare il sistema mettendo il *focus* sulla sostanza e non sulla forma, come purtroppo è adesso. Il coro di proteste che si è levato da parte di tutti gli operatori della giustizia la dice lunga su quali sono i rischi insiti in questa norma, non solo sul fronte delle garanzie per l'imputato, ma anche per quel che riguarda l'intasamento delle aule giudiziarie. La norma sull'agente di copertura andava definita con maggiore cautela. Qui, invece, assomiglia di più all'agente provocatore, ossia una figura che, anziché aiutare la magistratura a individuare i reati, provoca le persone a commetterne, ed è una deriva pericolosa del ruolo dello Stato e del rapporto che deve avere con i cittadini. E lasciano perplesse le norme sulla non punibilità per i corrotti che si pentono, così come quelle sulle pene accessorie, a cominciare da quella sull'interdizione perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che scatta automaticamente e priva il giudice di ogni possibilità di valutazione. Come con la legge sui permessi umanitari, con quella sulla legittima difesa e la famosa proposta Pillon, anche in questo caso si provano a introdurre nel nostro ordinamento norme-sentenza, che limitano la discrezionalità dei giudici di decidere caso per caso. Vi è poi tutto il capitolo che riguarda le norme sui partiti. Trovo significativo che queste norme vengano inserite in un provvedimento che voi definite spazza corrotti, quasi a voler suggerire all'opinione pubblica l'esistenza di una stretta correlazione tra politica e corruzione. Credo che questa continua svalutazione della politica sia una minaccia per la democrazia, anche perché, come si suol dire, la rivoluzione divorerà i propri figli. Quindi, basta con questa continua delegittimazione della politica alla quale appartenete anche voi. Prima o poi occorrerà fare una riflessione sui costi della politica, sulle forme del finanziamento, un tema su cui non c'è mai stata la serenità necessaria,

Come ha detto il senatore Balboni, domani direte che avete abolito i corrotti, come avete già abolito la povertà. E lo fate ponendo nuovamente la questione di fiducia, che congela il ruolo e le prerogative del Parlamento. I numeri, da questo punto di vista, cominciano a essere rilevanti: è la sesta volta che si ricorre a questo strumento, la seconda in Senato. Tutto questo non fa che accentuare il nostro giudizio negativo ed è per queste ragioni che il Gruppo Per le Autonomie voterà contro la fiducia.

come è noto, la corruzione è un reato senza testimoni, senza vittime, se non la collettività, e senza denunce, con un comune interesse degli autori al silenzio e all'omertà. La corruzione mina l'economia nel profondo, toglie trasparenza alle transazioni e agli appalti, privilegiando e favorendo i corruttori a danno degli onesti e dei più capaci. La corruzione disperde risorse, rallenta lo sviluppo, è tra le cause della mancata crescita economica. Senza contare i suoi costi indiretti, difficili da quantificare ma ugualmente rilevanti. Un terreno di coltura ideale perché la corruzione si diffonda e si trasformi in qualcosa di ancor più grave: l'accettazione che non vi siano alternative, la resa delle coscienze. Da procuratore nazionale antimafia chiedevo al legislatore l'inserimento del reato di corruzione tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, perché in questo modo avrebbero potuto usare tutti gli strumenti di contrasto previsti per il crimine organizzato. Avevo già da allora chiara la situazione sistemica e di stretta connessione, in certe Regioni italiane, tra organizzazioni criminali, potere politico, pubblica amministrazione e settori dell'economia e dell'imprenditoria. Si potrebbe dire, in sintesi, che ai mafiosi oggi convenga molto di più corrompere che sparare o intimidire; e le evidenze investigative lo dimostrano in maniera evidente. Dobbiamo tenerne conto. Un passo importante è stato compiuto, nella scorsa legislatura, con l'introduzione delle norme a difesa del *whistleblower*, cioè chi segnala un'irregolarità sul posto di lavoro. Ma con questo disegno di legge sull'anticorruzione si fanno, ebbene sì, due passi in avanti, a mio avviso. Il primo è la previsione di una causa speciale di non punibilità per chi denuncia. Ho ben Ho ben chiaro che il miglior risultato plausibile di questa norma sarà quello di insinuare un fattore di insicurezza che diminuisca la forza dell'accordo tra corruttore e corrotto: nessuna delle parti potrà più fare affidamento certo su un comune interesse a tacere e si determinerebbe quindi una sorta di deterrenza preventiva, un elemento che dissuada dall'entrare in un patto Il secondo è l'estensione ai reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui ho ampiamente parlato in discussione. Ricordo che nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono già previste per molti altri delitti, dalle estorsioni al sequestro di persona, dall'usura al riciclaggio, dai delitti contro la libertà sessuale al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal traffico di stupefacenti al traffico di rifiuti e - pensate - anche alla contraffazione di marchi e brevetti. *(Brusio)*. PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Grasso. Invito i colleghi che sono impegnati in conversazioni private a farlo con un tono di voce che non disturbi il senatore che sta intervenendo. Vi ringrazio. Se non parlassero sarebbe ancora meglio. PRESIDENTE. Sarebbe chiedere troppo. GRASSO *(Misto-LeU)*. Grazie per il tempo che mi farà recuperare. Non credo che la corruzione sia meno grave della contraffazione dei marchi. Si dice che questo istituto serva per i terroristi e che serva per i mafiosi. Non è vero: è stato già esteso a tutti questi reati dalla nostra legislazione vigente. La riforma della prescrizione andava inserita in un progetto organico di riforma del processo penale, che ora promettete di fare in pochi mesi. Io ricordo a tutti noi che, per riformare il processo, un insigne giurista come Giuliano Vassalli ci lavorò per dieci anni. Che ora voi ci mettiate dieci mesi, per una riforma, come voi dite, a 370 gradi, mi sembra onestamente difficile. Con rammarico, avendo voi messo la fiducia, non è stato nemmeno possibile discutere gli emendamenti che ho proposto come pacchetto tempi-giustizia. Del resto, a voi non interessa risolvere i problemi, ma avere medaglie di latta da esibire sui *social* e soprattutto prevenire ogni possibile dissenso che già forte serpeggia all'interno dei vostri Gruppi. Amici della maggioranza, a proposito di fiducia, ho letto che sulla vostra piattaforma Rousseau è stata inaugurata una pagina per le denunce e le delazioni contro quelli che tra di voi tradiscono i princìpi del MoVimento. Complimenti. Complimenti per l'idea di democrazia che state dimostrando. Lasciatemi fare allora la prima delazione, qui, pubblicamente: tutti voi, sia al Governo che in Parlamento, state tradendo quanto avete predicato per anni, nessuno escluso, né chi sta zitto e obbedisce, né chi rilascia dichiarazioni e interviste e poi si adegua, né chi critica, sempre a tempo scaduto, quando le decisioni sono state prese altrove. Sta diventando un'abitudine quella della fiducia; quando si inizia - è già successo ai vostri predecessori - è difficile smettere. In fondo, è molto più semplice costringere che convincere. Chiedetevi però quanto tempo potete durare, se già dopo pochi mesi ogni voto segreto vi terrorizza? Quanto a lungo pensate possano ancora funzionare le vostre finte liti sui giornali? Mi sembra invece una realtà che siete piuttosto uniti quando si tratta di occupare qualche poltrona. Quanto pensate che il gioco delle parti potrà durare,

Vale lo stesso per i colleghi leghisti. Oggi io, che sono a favore della sospensione della prescrizione e di quei rimedi per la corruzione, sarò obbligato a votare contro la fiducia al Governo, perché delle politiche di questo Governo non condivido praticamente nulla, a parte quello che ho appena detto. Voi invece, per contratto, voterete a favore. Non sentite l'ironia della cosa? Se non ricordo male, un vostro esponente, l'allora ministro Roberto Castelli, ricopriva l'incarico che oggi ricopre il ministro Bonafede, quando il Gruppo della Lega votò compattamente la legge ex Cirielli,

prendere nessuna iniziativa per accorciare i tempi del processo stesso. Questo significa votare la fiducia per voi: coprire con un obbligo ipocrita qualsiasi contorsione politica, rispetto agli ideali che avete sempre difeso e sostenuto. Su questi temi io non cambio idea, a differenza vostra. Avrei voluto discutere nel merito avrei voluto, a mio modo, aiutarvi a migliorare il testo. Alla fine, come ho dichiarato ieri su un quotidiano, avrei anche votato a favore, della fiducia e con l'impossibilità di intervenire, lo avete reso impossibile. Si tratta di un'altra occasione sprecata, a causa della vostra debolezza al Governo, nel Parlamento e presto - credetemi - nel Paese. Per questi motivi, con dispiacere,

*(PD)*. Signor Presidente, ci sono temi, in una democrazia, che chiamano all'impegno comune tutte le forze politiche e la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione è sicuramente uno di questi. Il Partito Democratico ne è sempre stato convinto, in questo senso ha sempre lavorato e lo ha fatto anche sul provvedimento in esame, nonostante il silenzio assordante e imbarazzante delle

che saranno chiamate a toccare con mano il prezzo assurdo della vostra propaganda. Lo possiamo fare anche perché, non da oggi, siamo convinti che la prima vittima della corruzione sia proprio la buona politica. Se nella pubblica amministrazione avanza l'illegalità è la politica a diventare meno efficace, credibile ed autorevole ed è la sua capacità di decisione e di intervento a diventare sicuramente meno efficace. Il nostro sarà un voto convintamente contrario al disegno di legge in esame e alla questione di fiducia. Sarà un voto contrario per l'impianto culturale del provvedimento in esame, che è profondamente antidemocratico e illiberale, un voto contrario per gli scarsi risultati che si perseguono con le scelte compiute, ma anche e soprattutto un voto contrario per il prezzo mostruoso, in termini di garanzie, di diritti e di spazi di libertà che viene imposto in nome di una semplice e presunta lotta alla corruzione. Di lotta alla corruzione vera ed effettiva, infatti, all'interno del provvedimento in esame ce n'è davvero poca. Per questo nessuna manifestazione di piazza, nessun tono enfatico, nessun annuncio pirotecnico riuscirà a coprire i vuoti e l'inefficacia di questo provvedimento che mostra soltanto la distanza abissale che passa tra i vostri annunci e gli atti di governo. Oggi abbiamo la dimostrazione che il vostro patto di potere - quello che voi chiamate contratto - si regge sullo scambio di un reciproco interesse: a un pezzo di voi campo libero per cavalcare e usare a proprio uso e consumo le paure di chi chiede più sicurezza; campo libero per cavalcare nella stessa maniera la rabbia di chi chiede una politica più onesta e trasparente. Ma c'è di più. Nel "decreto insicurezza" avete abbinato il tema della sicurezza a quello dell'immigrazione; al tema della corruzione collegate la trasparenza dei partiti. Lo fate con un messaggio recondito, ma insieme chiaro e pericoloso: l'insicurezza la portano gli immigrati, la corruzione i partiti. intestandovi una strategia pericolosa per il tessuto democratico e la salvaguardia di uno stato di diritto, e tutto solo per venire qui in Aula e davanti al Paese a recitare la parte dei moralizzatori. Ci dispiace svegliarvi da questo bel sogno e riportarvi con i piedi a terra: su questo terreno siete fuori tempo massimo; per questo copione non siete più credibili. A nessuno in quest'Assemblea compete il ruolo di pubblico ministero dell'etica pubblica, ma soprattutto a nessuno di voi questo ruolo sarebbe consentito, men che meno a coloro che siedono tra i banchi del Governo. Provo a ricordare a noi tutti, non siete forse voi quelli che hanno sdoganato odiosi condoni ergendosi a paladini di una delle forme di illegalità

Che credibilità può avere chi sa sa che la prima alleanza da fare per combattere la corruzione è quella con magistrati e Forze dell'ordine, e ogni giorno da questo Governo arrivano attacchi che minano la credibilità della magistratura senza che lei, ministro Bonafede, alzi mai la voce a difendere quella magistratura? ve la consentiamo. Non ve la consentiamo proprio perché la lotta alla corruzione è un problema serio, vero, da affrontare con rigore e serietà. Del resto, nessuna sorpresa; almeno vi va riconosciuta una coerenza nella sceneggiatura. Li ricordiamo tutti i vostri voti e le vostre parole quando su questo terreno abbiamo cercato di fare qualcosa di serio. Lo hanno già ricordato i miei colleghi quindi procedo spedita: le pene per reati contro la pubblica amministrazione, il falso in bilancio, la sospensione condizionale della pena, il ruolo dell'ANAC. Ricordiamo i vostri voti, ricordiamo i vostri commenti. Eppure noi, oggi dall'opposizione eravamo pronti anche a migliorare quegli interventi perché non abbiamo la presunzione - a differenza vostra - di dire «dopo di noi, il diluvio». Sappiamo che la lotta alla corruzione richiede un impegno continuo, su più livelli: che non si abbassi mai la guardia della risposta repressiva ma che, soprattutto, si diano strumenti di prevenzione più ampi. Per questo oggi la scelta da fare, signor Ministro, cari colleghi della maggioranza, richiedeva coraggio, serietà e rigore, caratteristiche del tutto assenti nella vostra maggioranza. Proseguire nella riforma della pubblica amministrazione, aumentare la qualità del servizio offerto in primo luogo attraverso percorsi di semplificazione organizzativa e trasparenza dei procedimenti: era questa la scommessa da vincere. Da qui passa la legalità dei comportamenti. Solo così si rende la pubblica amministrazione impermeabile a fenomeni corruttivi. Me ne rendo conto, è una strada per voi lunga e faticosa, ma è l'unica possibile per fare sul serio. Voi ne avete scelto un'altra: quella basata solo e soltanto sulla repressione dei fenomeni criminali. La vostra è la strada più facile; purtroppo però per il Paese e per gli italiani, anche quella meno efficace e insieme più pericolosa. Dite di voler rendere precario l'accordo correttivo, e inserite l'agente sotto copertura e la causa di non punibilità. Avete voluto alzare il tiro. Avete detto: se non si può mettere l'agente provocatore, con la causa di non punibilità sostanzialmente lo inseriamo ugualmente. Abbiamo cercato di migliorare questo testo e anche in questo caso vi abbiamo ricordato la vostra incoerenza. Riconoscete con belle parole il lavoro e il merito del presidente dell'Autorità nazionale

giustamente invocate, si realizzi non a scapito di diritti e garanzie sacrosanti dei cittadini, ma facendo leva su una macchina giudiziaria dotata di strumenti investigativi forti, ed anche, soprattutto, di maggiori strumenti e risorse organizzative e strumentali per i nostri uffici giudiziari. Quelle voci che voi avete ignorato in queste settimane non ci chiedevano più tempo per arrivare a sentenza, ma più risorse per arrivarci in meno tempo e in maniera più efficace, incisiva e, soprattutto, giusta. Dopo un mese e più di discussione, nessuno ha ancora capito in quale modo lo *stop* alla prescrizione dovrebbe favorire la ragionevole durata dei processi. La conseguenza è che ci saranno processi infiniti e imputati colpevoli a prescindere, cui far pagare la sofferenza del processo prima che intervenga una sentenza definitiva. Sbaglia chi pensa che la vostra sia stata una scelta inconsapevole. È stata un'operazione cinica e pericolosa perché avete scelto di scaricare i costi del nostro sistema giudiziario sui cittadini, su coloro che - innocenti o colpevoli non importa - entreranno nel *tunnel* del processo e non sapranno quando ne usciranno, dando così il benservito a uno dei princìpi cardine del nostro ordinamento: la ragionevole durata del processo.

le sue tesi d'accusa in un tempo ragionevole e che rinuncia perciò - e soltanto per questa ragione - alla sua pretesa punitiva verso un presunto innocente. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ripeto: nel nostro ordinamento vale il principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Sulla prescrizione avete scelto deliberatamente di non guardare i dati della normativa attuale su uso delle pene accessorie, innalzamento dei massimi di pena e non punibilità. Avete fatto norme a efficacia minima, ma a pericolo massimo. Fate come se logica e strumenti usati per la lotta alla grande criminalità organizzata e al terrorismo possano applicarsi automaticamente alla lotta per la corruzione, quella grande e meno grande, ma molti pubblici ministeri che avete audito vi hanno detto che non è così (e voi sapete che non è così). Penso, in particolare, alle deroghe che prevedete per l'uso del *trojan*, uno tra gli strumenti investigativi più invasivi

Non è un caso che uno dei primi atti di questo Governo sia stato il buttare a mare la riforma penitenziaria, riproponendo così l'idea che il carcere sia l'unico strumento utile per punire e reprimere il crimine. Su questo tra 5 Stelle e Lega la comunione di intenti è massima, altro che divisione! Voi vi fregiate del fare le leggi con il solo scopo di rispondere alle richieste dei cittadini. Non vi rendete conto che il rischio è di esercitare la giustizia con il pollice verso. Questa però non è più giustizia, ma arbitrio, non è presunzione di innocenza, ma sospetto di colpevolezza per tutti.

e di una cultura giuridica, che il mondo intero ci invidia, il Partito Democratico ci sarà sempre. In compenso, la vera lotta alla corruzione la rimandate a non so quando e con essa rinviate *sine die* la battaglia per un'amministrazione efficiente e trasparente, così come quella per una buona politica. Ma noi non ci arrendiamo: continueremo a lavorare per arginare i danni delle vostre scelte irresponsabili e propagandistiche e per fare in modo che tra i cittadini la giusta richiesta di una buona politica e di una buona amministrazione impermeabile ai fenomeni corruttivi divenga sempre più lontana da propaganda e demagogia e sempre più vicina a una politica seria, rigorosa e per questo efficace e concreta. Per queste ragioni il nostro sarà un voto orgogliosamente e convintamente contrario a questo provvedimento e, soprattutto, a questo Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in premessa devo dare atto della coerenza del Partito Democratico che, come sempre gli capita quando non sa che dire, divaga.

ai colleghi del Partito democratico che appartengono a quella cultura politica che, con la legge Severino, ha accorciato i termini di prescrizione per aiutare il portaborse del loro ex segretario di partito. Potrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che appartengono a quella cultura politica che in una notte d'estate ha abolito l'abuso d'ufficio per aiutare

Vorrei ricordare, Presidente, che quella cultura politica, in un frangente di questa Repubblica, ha addirittura provato ad aiutare Sofri, Bompressi e Pietrostefani,

caro Ministro, spero che il presidente Bolsonaro finalmente assicuri Battisti alle patrie galere per i crimini schifosi che ha commesso qui in Italia.

partendo da un assunto: il fenomeno corruttivo, purtroppo, è radicato ed è diffuso nella politica e nella pubblica amministrazione italiana. Pertanto è un fenomeno che va spazzato via con una legge importante. Tra le tante cose che ho sentito durante questo dibattito (alcune coerenti rispetto al provvedimento, altre meno), non ho sentito parlare dell'effetto deterrente della norma penale. È un effetto

per dire ai cittadini «basta commettere determinati reati». Noi parliamo, come ha detto il senatore Grasso, di reati che hanno un impatto sociale pesantissimo. Infatti, la parte offesa di questi reati è l'opinione pubblica e la comunità nazionale o può essere una comunità cittadina: di questo parla il disegno di legge anticorruzione. Non parla di quanto ho anche sentito dire, cioè di delitti colposi. Qualcuno faceva accenno alla responsabilità dei sindaci, per esempio, nelle lesioni colpose o negli omicidi colposi, ma questo non esiste. Così come non esiste all'interno di questo provvedimento l'abuso d'ufficio, che è la tagliola in cui tutti quanti gli amministratori comunali (lo dico anche da sindaco) rischiano di incappare in maniera più frequente. Questo è un reato che all'interno del provvedimento non è assolutamente annoverato. Un'altra riflessione vorrei farla rispetto al giusto processo e vorrei farmi e fare a questa Assemblea alcune domande: il processo attuale è un processo giusto, sì o no?

in una ragionevole durata, sì o no? È un processo che nella fase delle indagini viene condotto in maniera riservata, sì o no? o no? Partendo dalla prescrizione, pochi hanno rilevato che è un istituto che avrà efficacia contestualmente all'avvio del nuovo processo penale, ovvero dal primo gennaio 2020. Ritengo allora che questa sia la sfida più importante; fare un processo che assicuri trasparenza, parità effettiva tra accusa e difesa e, soprattutto, celerità. Se infatti un processo si celebra con celerità, viene garantito lo Stato assicurando la pena al colpevole, ma soprattutto viene garantito l'innocente, che non è costretto a subire

La vera sfida è allora quella del nuovo procedimento penale. Una norma va vista nella sua praticabilità e nei suoi effetti rispetto al processo penale. Questa è la sfida che il Governo ha accettato

la libertà è un valore irrinunciabile: la nostra, ma soprattutto, per certi versi, quella degli altri. Qualcuno amava definirla come l'ossigeno: senza non si vive. Ricordo che la libertà non si decanta, ma si conquista e si difende. In passato i nostri padri l'hanno fatto con atti eroici, a noi spetta farlo con atti di civiltà e quest'atto può essere il nuovo processo penale che la legge delega assegnerà al Governo.

mi verrebbe da dire «benvenuti sulla terra». Signor Ministro, parlo con lei. Mi sembra infatti che voi eravate quelli che vi opponevate ai Governi che mettevano la fiducia; eravate quelli che occupavate i banchi del Governo per protestare contro gli atti che limitavano la libertà e la libera coscienza dei parlamentari. Oggi, invece, ponete la fiducia proprio per controllare i vostri parlamentari

che c'entra la prescrizione? Essa era stata già regolata un anno fa dal ministro Orlando, dal Governo di centrosinistra che l'aveva aumentata

Il collega che mi ha preceduto parlava di un processo giusto in tempi rapidi, voi lo allungate e lo ritenete ingiusto, creando una disparità di trattamento tra accusa e difesa!

mi dai l'anticorruzione e la prescrizione, io ti do la sicurezza. Un Paese non può però fondarsi su questi patti.

finirà la pacchia degli avvocati azzeccagarbugli che con i loro espedienti allungano il processo. Ministro, lei forse non sa che dal 2001 i rinvii chiesti dall'avvocato e dall'imputato sospendono automaticamente la prescrizione. Altro che azzeccagarbugli! Lei allunga la prescrizione, violando l'articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo e l'articolo 6 della Convezione per la

vent'anni: come fa a giustificare la ragionevole durata del processo? E la legge Pinto? Lei sta creando un varco nel quale lo Stato sarà costretto a pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento danni per la irragionevole durata del processo. Le dico anche una cosa, che forse le sembrerà strana: con questa legge, lei raggiunge esattamente l'effetto opposto a quello che si è prefissato; lei con questa legge vuole spazzare la società da corrotti e corruttori e invece li agevola, perché se allunga fino a vent'anni i tempi della prescrizione, consente a costoro di continuare a commettere reati per vent'anni, altro che spazzare via dalla società i corrotti! Lei sa, signor Ministro, che nel nostro Paese ogni anno 7.000 cittadini vengono dichiarati non colpevoli dopo aver patito la carcerazione preventiva? Lei sa che un terzo dei processi si conclude con una sentenza di assoluzione? A lei è mai capitato di difendere o di venire a conoscenza di situazioni di amministratori locali che sono stati buttati in carcere, che sono stati indicati al pubblico ludibrio, che sono stati distrutti nella carriera, negli affetti, nella famiglia, nella dignità e sono stati assolti dopo dieci anni, quando ormai non avevano più bisogno neanche delle scuse dello Stato? Lei ha un merito: vuole introdurre nel nostro ordinamento il processo eterno. Noi pensavamo che ci fosse la vita eterna: lei ci insegna, con questo provvedimento, che c'è il processo eterno. La ringraziamo.

parliamo di giuristi illuminati, voi oggi siete più interessati a contendervi i *like* sui vostri profili piuttosto che a rispondere alle esigenze del Paese. Questa norma, però, viola anche l'articolo 27 della Costituzione, perché sostituisce alla presunzione di innocenza quella di colpevolezza. Signor Ministro, non so lei che concetto abbia del processo, ma il processo non è un luogo dove il colpevole cerca di farla franca: molto spesso è una tragedia che si abbatte su un cittadino al quale viene riconosciuta l'innocenza quando ormai è stato distrutto in tutti i suoi valori. Dove è finito il principio costituzionale della rieducazione della pena? Che senso ha condannare una persona dopo quindici o vent'anni dal commesso reato? La persona che espierebbe la pena è una persona completamente diversa da quella che commise il reato.

è una norma a favore delle parti lese, perché non ci saranno più prescrizioni, e ha citato l'esempio del disastro di Viareggio. Mi verrebbe da dire che lei ha detto una fesseria, ma per rispetto istituzionale dico che lei ha detto un'inesattezza.

Avete inserito i reati contro la pubblica amministrazione paragonandoli a quelli mafiosi. Avete introdotto la possibilità di utilizzare l'agente sotto copertura,

che non sa difendere i cittadini. Avete ridotto l'accesso ai benefici penitenziari e state creando le condizioni per far saltare il sistema detentivo, già al limite; aumentate le pene e limitate l'accesso alle misure alternative, ma quando varerete un piano di edilizia penitenziaria e di arruolamento di polizia penitenziaria? Fate la faccia feroce, ma scaricate le vostre inadempienze sul sistema!

Complimenti, avete fatto esattamente il contrario: autorizzare l'accesso indiscriminato alle banche dati e ai conti correnti dei contribuenti, senza il controllo dell'autorità giudiziaria, e prevedere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, anche in caso di sospensione della pena, fanno sì che il cittadino sia visto sempre con pregiudizio dallo Stato. Non avete fiducia neanche nella magistratura, che dite di vantare e tutelare. Avete sottratto al giudice la possibilità di graduare l'entità e la durata della pena accessoria in base alla gravità dei fatti e sulla base del suo prudente apprezzamento. Oltre a violare esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, avete inciso sul principio della proporzionalità. Se di riforma si doveva parlare, non potevate cominciare peggio, intervenendo sul processo al contrario, senza diminuirne i tempi, ma allungandoli. Mi rivolgo agli amici della Lega, con i quali abbiamo votato la riforma sulla prescrizione, la cosiddetta ex Cirielli, abbiamo introdotto in maniera stabile l'articolo 41-*bis*, 41-*bis*, abbiamo modificato tutta la normativa antimafia e abbiamo aumentato le pene per i reati nella pubblica amministrazione: come fate a votare un provvedimento di questo tipo? *(Applausi State creando un mostro giuridico, del quale voi stessi sarete vittime, ma questo ci interessa poco, perché chi è artefice del proprio destino pianga se stesso; purtroppo, però, ne saranno vittima i cittadini, anche quelli che vi hanno votato

decreto sicurezza, che è un topolino partorito da una montagna; il provvedimento sulla concretezza, che, al contrario, crea ostacoli e anziché sburocratizzare aumenta le problematiche; il decreto anticorrotti, che invece di reprimere il fenomeno lo incoraggia. Vi Vi invito a fermarvi finché potete e soprattutto a cercare, per il tempo che vi resta, di non fare più danni di quelli che potremo umanamente riparare quando - e quel tempo è molto vicino torneremo a governare questo Paese. Per tali ragioni, voteremo convintamente contro la fiducia a questo provvedimento.

il provvedimento di legge che stiamo per approvare merita grande rispetto e considerazione. Ho ascoltato cose che

lunghissimo, senza che sia stato affrontato il problema con il dovuto coraggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. C'è stato qualcuno che, nel 2015, visitando il quartiere di Scampia, zona famosa per camorra e non per corruzione, ha detto che la corruzione è il linguaggio di cui si servono le mafie per corrompere i pubblici ufficiali. Questo qualcuno era Bergoglio, il pontefice che voi citate molto spesso,

Quando Bergoglio sostiene che la corruzione spuzza, tutti quanti ad applaudire e ad osannarlo, Presidente. Quando poi, però, bisogna perseguire comportamenti contrassegnati appunto da volontà corruttiva o comunque di accettazione di tale volontà,

colpito le pubbliche amministrazioni e le classi dirigenti delle stesse pubbliche amministrazioni, senza che siano stati mai perseguiti veramente. Senza allora voler tornare allo scandalo della Banca romana,

noi abbiamo necessità di un provvedimento che quantomeno indichi che questo Stato sta cambiando, il termine giusto che vorrei uscisse da queste Aule è «cambiamento».

la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente possa essere inutile

e pretende anche una sorta di coraggio che molto spesso alcuni singoli non si riconoscono. della corruzione», che dovrebbero farci riflettere tutti: «In vita mia non avevo mai visto un corrotto. Me l'immaginavo come un *visitor,* con la lingua verde che fuoriesce dalla bocca, e quando le guardie mi portarono questo detenuto rimasi impressionato dalla sua assoluta normalità». Qualcuno potrebbe anche ricordarsi Hannah Arendt, perché quello che ci deve colpire è «la banalità del male» e, pertanto, la normalità della corruzione. «Era uno come me. Avrebbe potuto essere un mio compagno di università o di serate in discoteca. Allora misi via il foglietto con gli appunti e l'unica domanda che formulai fu: "Ma come può un ragazzo di ventisette anni vendersi per 250.000 lire?". L'imputato per un po' rimase in silenzio e poi rispose: "Lei non può capire, perché appartiene ad un mondo del quale queste scelte sono soltanto individuali: essere onesto o disonesto dipende da lei. Io, dopo quindici giorni dal mio arrivo, ho capito che in quell'ufficio" - un ufficio pubblico - "rubavano tutti! E ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di un uomo onesto." - perché l'onestà non può essere ammessa "Mi avrebbero cacciato perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Le 250.000 lire me le ha messe in mano il mio capoufficio. Io ero in prova, e ho avuto paura di essere cacciato via se non le avessi prese.

purché tutto sia secondo norma, a chi la vuole farla finita con un certo mondo per cui la disonestà è il modello, di poterla far finita e quindi di passare dal crimine allo Stato. Aggiungo anche Aggiungo anche che proprio pochi giorni fa hanno consegnato le motivazioni per la sentenza in appello della vicenda

l'intimidazione, che è tipica del comportamento mafioso, e qualcun altro (Buzzi) ci metteva la corruttela, cioè la propensione ad acquistare assenso da parte di pubblici amministratori, di pubblici ufficiali che dovrebbero rappresentare lo Stato ma che si svendono per soddisfare loro egoistici interessi, danneggiando lo Stato tutto e soprattutto i più deboli! *(Applausi Badate che accettare una bustarella (perché così si inizia) equivale ad accettare con mano il comportamento di chi si presenta con la lupara in spalla. Accettare la bustarella significa impedire che in una terra che vive oggi in molta parte della sua popolazione il dramma, la tragedia della miseria, si possa far spesa sociale, perché se si permette al privato indebitamente di frodare lo Stato, non solo si sta frodando lo Stato, si sta frodando il più debole dei cittadini di quello Stato. Pertanto, chi combatte la corruzione lo fa per i valori della democrazia e non di altro e questo voi non lo avete mai praticato *(Applausi dal Gruppo

si salvaguarda anche - e questo abbiamo fatto nella norma - non soltanto aumentando i massimi edittali della pena, ma soprattutto elevando i minimi di pena.

tanto più le pene erano inferiori al passato, quasi a voler dire: «Vabbè, lo facciamo tutti, quindi indulgenza plenaria per corrotti e corruttori». Questo non va

saranno contentissimi nel sapere che, finalmente, chi froda lo Stato avrà difficoltà a continuare a contrattare con lo Stato e a rappresentare lo Stato. Chi è uomo di Stato ha una dignità enorme e anche nel più umile dei servitori dello Stato vi deve essere quella disciplina, quell'onore che fa sì che lavorando per lo Stato - e cioè per noi tutti - non si accetti alcuna pratica corruttiva, non si metta in atto alcun comportamento criminale, paramafioso, che affossa la democrazia. Le interdittive temporanee per chi incorre in pene inferiori a due anni (ma anche e soprattutto definitive) sono allora ciò che tutti i cittadini onesti vogliono, perché non possiamo più consentire che lo Stato sia il bancomat presso cui tutti quanti prelevano senza aver precedentemente depositato!

Regione Calabria la dirigente responsabile dell'anticorruzione è stata anche lei arrestata per corruzione. *dal Gruppo FI-BP)*. Se allora noi accettiamo che nei territori più deboli, lì dove vi deve essere ancor più vigilanza, ancor più controllo, ancor più trasparenza,

so che ragionare di onestà dà problemi a tanti, però io penso che a tutti quanti gli italiani farebbe piacere il rovesciamento di quella frase tristissima, che è riportata nel testo di Piercamillo Davigo da cui ho attinto: noi non dobbiamo essere il Paese in cui c'è necessità di coraggio per essere onesti; noi dobbiamo essere il Paese in cui, con fierezza, si deve essere onesti!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

senatore Parrini).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Parrini.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Signor Presidente, intervengo in merito ai fatti di Strasburgo dell'altro giorno. La gravità di quanto accaduto non necessita di ulteriori note. note. Colleghi, voglio farvi ricordare quanti minuti di silenzio si siano svolti: a quanti minuti di silenzio avete assistito? Quante dichiarazioni di cordoglio, quanti «Mai più»? Ricordate i gessetti colorati? Conoscete la gravità dell'evento che è successo e anzitutto mi unisco alla solidarietà verso la famiglia di Antonio Megalizzi, il nostro connazionale attualmente in condizioni disperate in ospedale. Il luogo che è stato colpito è il mercatino di Natale presso la cattedrale di Strasburgo. Questo mercatino risale al 1570, è una tradizione che attiene alle nostre radici più profonde, quelle radici cristiane

già noto alle Forze dell'ordine per posizioni estreme, ha una caratteristica in comune con i colpevoli di mille altri eventi occorsi in Europa e nel mondo, ovvero la sua visione del mondo, la sua ideologia e la sua religione: è un musulmano. Vi posso dire che uno dei primi comunicati stampa delle Agenzie europee nelle ore immediatamente successive all'evento è stato fatto dalla dalla comunità islamica locale di Strasburgo, che con tragicomico cinismo ha affermato che le vere vittime di questo attentato sono i musulmani. Spieghiamo bene: si spara per le strade, si uccidono cittadini europei e non solo europei e gli occidentali, che tollerano queste comunità poco tolleranti nei nostri confronti, sono colpevoli, a prescindere, di razzismo. Guai a ribellarsi al fatto di essere bersagli di un attentato! Tant'è vero che

Rousseau, ma l'ha detta Gesù Cristo ed è riportata nel Nuovo Testamento, per noi è un principio scontato, perché connaturato alla nostra religione ed è scontato perché è connaturato ai principi della democrazia. attenzione, perché questi princìpi sono molto delicati e c'è da chiedersi - concludo, signor Presidente - se l'Islam è integrabile nella nostra democrazia. Questa ideologia - e non religione - lo è? Per me no e con questo concludo e vi invito a riflettere.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

La seduta è tolta